L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Signora Presidente, il provvedimento in esame ci richiama ad una responsabilità molto grande che ha davanti il nostro Paese per restituire credibilità alla politica, alle istituzioni, per promuovere una riforma fondamentale di tanti assetti di questo Paese, dalla pubblica amministrazione al sistema giudiziario, per favorire la crescita di un'etica e di una responsabilità che coniughi serietà, rigore e sobrietà. Il fenomeno corruttivo, che è in costante crescita in Italia, così come ci indica la Corte dei conti nelle sue analisi, dimostra che molto di questo malaffare si insedia e si annida dentro le pubbliche amministrazioni e che questo elemento rappresenta la quarta fonte di danno erariale in ordine di importanza. L'espansione del delitto e del fenomeno corruttivo sicuramente anche strettamente connessa ad una percezione che nella collettività è diventata sempre più bassa rispetto al disvalore di tali reati e alla loro incidenza sulla gestione della cosa pubblica.

Le azioni che dobbiamo mettere in atto sono, oltre la promozione di una etica pubblica e di una cultura diffusa della legalità, anche quelle specifiche attinenti al funzionamento della pubblica amministrazione, alla trasparenza, al tema degli appalti e al contrasto di detto fenomeno nel pubblico come nel privato. È per questo che ci chiediamo, almeno sul versante pubblico: dove è la tanto declamata riforma della pubblica amministrazione? Dove è la riforma del ministro Brunetta? Si potrebbe dire «Chi l'ha vista?». Nel maggio 2008 il Ministro lanciava un grande piano industriale con linee programmatiche sulla riforma della pubblica amministrazione, per porre al centro il merito, la produttività, l'efficienza e la trasparenza. Abbiamo convenuto e contribuito anche alla costruzione della legge delega con le nostre proposte e i nostri emendamenti per mettere al centro la valutazione, la trasparenza, l'integrità della pubblica amministrazione e per favorire un organismo indipendente che svolgesse tale compito. Gli intendimenti del Ministro sono stati - dobbiamo dirlo - soltanto fumo: qualche trovata pubblicitaria come le "faccette con il sorriso" per introdurre la valutazione da parte degli utenti; nessun costrutto per avviare una riforma seria e aprire un cantiere profondo all'interno della pubblica amministrazione, centrale e periferica. Forse non si poteva farlo, visto che in quei tempi e in quei momenti si andavano sviluppando fenomeni corruttivi che hanno interessato anche la gestione di questo Governo. Il primo *report* di Cittadinanzattiva sui dati 2009 ci dice che la trasparenza non c'è, e si vede; che i cittadini denunciano situazioni di opacità per mancanza di informazioni

con paurosi ritorni indietro. Dove sono i controlli sulle prestazioni erogate, la lotta agli sprechi, la valutazione che premia il merito, i meccanismi che avrebbero dovuto consentire il controllo sui servizi pubblici, la "responsività" come capacità di rendere conto di scelte e comportamenti agli interlocutori delle pubbliche amministrazioni? Dove è il grande cantiere che si doveva e si dovrebbe aprire? Le nostre proposte si muovono su questo terreno, per dare efficienza e produttività alla pubblica amministrazione, per migliorare la sua capacità di azione, per illuminare gli angoli bui in cui si annida la corruzione. Tutto si deve conoscere: nomi, incarichi, compensi, appalti, la loro storia, la loro vita, il loro procedimento, per consentire controlli incrociati sulle forniture, sui compensi e su quant'altro connesso. Il cittadino deve essere coinvolto nella valutazione della prestazione dei servizi, perché questo determina possibilità di maggiore trasparenza. Bisogna rimuovere tutte le possibilità di cumuli di incarichi, di sovrapposizioni di funzioni tra controllori e controllati e i conflitti di interesse espressi e potenziali. Una agenda di riforme mancate, quindi, di cui dovrete dare spiegazioni al Paese, alle imprese, ai cittadini, ai giovani. E ancora, con questo disegno di legge, che abbiamo molto voluto e richiesto, troviamo passi indietro e sicuramente mancate risposte. Che cosa dire del sistema degli appalti su cui varie forme di prevenzione e di controllo sarebbero fondamentali, i patti di integrità da inserire nei bandi di gara per favorire i controlli incrociati, la qualità e la concorrenza? L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici rispetto a lavori e servizi come sia necessario che la banca dati dei contratti pubblici acquisisca altri dati di interesse al fine di costituire un'unica banca dati di controllo, per includere modalità nuove di acquisizione, per far sì che si costituisca una anagrafe unica, affinché essa possa essere interoperativa con l'anagrafe tributaria, con il casellario giudiziario, con la Direzione nazionale antimafia, indipendentemente dall'importo, dalle modalità di aggiudicazione, anche per i contratti in deroga; prevedere l'obbligatorietà del codice identificativo del contratto e - come indicato dall'OCSE - fare molta attenzione alle zone grigie della vulnerabilità delle gare, sia prima che dopo, nelle forme di evidenza nei pagamenti. La corruzione è un fenomeno che ha un impatto economico nel nostro Paese calcolato intorno ai 60 milioni di euro. Pensate: 1.000 euro l'anno per ogni bambino nato. È un costo questo che non ci possiamo permettere, permettere, che non ha solo a che fare con l'etica pubblica ma anche con la competitività del nostro Paese, con la possibilità di crescita, con il futuro delle giovani generazioni. Ha a che fare con la modernizzazione e l'innovazione dell'Italia, che ha bisogno di essere tale per potere competere. La maggior parte dei reati di corruzione si consuma nelle pubbliche amministrazioni e mentre questo prima era considerato un fenomeno marginale di alcune aree del Paese, oggi si vede come i fenomeni corruttivi si estendano, si confondano, si intreccino alla criminalità organizzata, vadano da Nord a Sud e riguardino funzionari pubblici, imprenditori, professionisti, rappresentanti politici e istituzionali. Occorre quindi darci strumenti sofisticati e qualificati, cosa che non ritroviamo in questa proposta di legge, che ci sembra, a dir la verità, per molti aspetti deludente. Queste sono le nostre proposte, questi i nostri contributi. Abbiamo tanto lavorato perché la Commissione sulla pubblica amministrazione e la trasparenza fosse attiva; in realtà è lasciata a se stessa, priva di risorse, un po' sul binario morto. La corruzione deteriora la pubblica amministrazione, è un ostacolo al corretto funzionamento del mercato, su cui occorre invece ricercare il miglioramento, l'innovazione, la crescita complessiva dei fattori di competitività. È per questo che insistiamo ed abbiamo insistito molto su questo provvedimento, perché esso fosse serio, profondo e andasse alla radice di tanti problemi. Ma questi temi possono sembrare, nel clima politico e nel panorama istituzionale, forse, per l'immagine che sta dando questo Paese anche all'estero, quasi risibili e perfino incredibili, forse in controtendenza. E non basta una operazione di facciata: vedremo nel corso dell'analisi di questo provvedimento se le nostre proposte saranno prese in considerazione, e come ho già detto, se alcuni degli stralci, che ci paiono a dir la verità davvero pericolosi e sicuramente un passo indietro rispetto allo stesso testo, saranno portati avanti. Noi vogliamo condurre una battaglia per parlare all'inquietudine, alla sfiducia, alla stanchezza, alla assuefazione di tanti cittadini onesti che accrescono la loro distanza verso la pubblica amministrazione e le istituzioni. Vogliamo restituire con proposte concrete, con serietà, con rigore, speranza e fiducia per una stagione nuova, nell'interesse del nostro Paese e per le nostre future generazioni.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, stamattina diciamo «onorevoli colleghi», se fossimo intervenuti ieri sera avremmo detto «onorevoli banchi», perché non c'era più nessuno. quindi un onore ed una opportunità quella di intervenire da ultimo in discussione generale stamattina e, poiché ho ascoltato disciplinatamente e diligentemente tutti gli interventi, con particolare riferimento a quelli dei colleghi dell'opposizione di sinistra, non voglio privarmi del piacere di rendere a braccio qualche considerazione, ancorché un po' politicamente poco corretta, come mi è abituale. La prima considerazione è che ho sentito invocare dei banchi di sinistra, reiteratamente, «una nuova *Authority*», «una Autorità indipendente», «veramente indipendente», la «costituzione di una nuova Autorità». Ora, ricordo che un paio di legislature fa avevo l'onore di presiedere a Montecitorio la Commissione lavoro ed arrivò una proposta per la istituzione di un Alto commissariato per la repressione del malcostume e della corruttela nella pubblica amministrazione, con un titolo lungo tre righe. Per la verità, ancorché esponente, forse anche non di ultimissima linea, della maggioranza, dissi che non volevo votare quella proposta perché, essendo un po' all'antica, mi chiedevo: mi chiedevo: ma è possibile che in un Paese civile si debba istituire una autorità, un alto commissariato per verificare che non ci sia corruttela nei gangli della pubblica amministrazione? Mi ricordo che fui anche un po' blasfemo, perché dissi: «Scusate il paradosso poco riguardoso, ma sarebbe come se l'autorità ecclesiastica dovesse istituire un alto commissariato per verificare che nei monasteri non si pratichi droga e prostituzione!». Non lo capisco. Sarò ottocentesco, sarò della destra storica, sarò quel che vi pare, fatto sta che non concepisco che si debba mettere in piedi un organismo con 50 o 100 dipendenti per monitorare i funzionari pubblici e i loro capi ufficio, che hanno come primo dovere, fino a prova contraria, quello di controllare che non ci sia malcostume nei propri uffici, negli uffici da loro diretti. ci dovesse essere un altro organismo, un'altra farragine sopra, pagata naturalmente dal contribuente, per verificare che non ci fossero deviazioni e malcostumi. Allora, anche su questa storia del mettere in piedi nuovi organismi personalmente non sono d'accordo,

o comunque debbono avere una valutazione professionale infima e censuratrice, che li deve escomiare dai loro incarichi. Quanto poi agli accenti, credo sinceri da parte della grande maggioranza di coloro che hanno parlato, usati riguardo al fenomeno del malcostume, della corruttela, dei profitti nella pubblica amministrazione,

alla Toscana e all'Emilia Romagna, non facciamo altro che leggere paginoni di interviste ad esponenti della sinistra e del Partito Democratico, e in particolare anche a parlamentari autorevolissimi, che fustigano il loro stesso partito dicendo che c'è una grave questione morale da affrontare, che va ben al di là della questione giudiziaria che, all'insegna dei casi di «sanitopoli», «amministrativopoli» e «regionopoli», si sta intrecciando in quel santuario del potere della sinistra appenninica. Ormai questo è diventato il Partito Democratico insieme ai suoi alleati: una roccaforte di potere e sottopotere appenninico e centro-italiano. Questi autorevoli esponenti sono forse traditori del loro partito? Assolutamente no: non mi sento di dirlo, e non penso che nessun osservatore oggettivo e intelligente lo direbbe. Questa è invece la denunzia di un fatto gravissimo e consolidato nella tradizione della sinistra di potere in intere zone del nostro Paese, in cui non c'era un'assicurazione comunale che non andasse in una certa direzione, né un concorso: si spartivano anche l'ultimo bidello, in una maniera scientifica. Non c'era famiglia che non percepisse indebitamente quello che non doveva percepire. Non c'era particella del piano regolatore che non venisse dichiarata edificabile o non edificabile a seconda di chi ne fosse proprietario. Non c'era situazione in cui, mentre una famiglia bisognosa

nessuno è vergine e nessuno è immune, ma che si vengano a usare certi accenti o certi toni particolarmente sdegnati rispetto a una situazione di potere, di sottopotere, di corruttela e di favoritismo, che largamente è stata perpetrata e consolidata da certe forze politiche, è una cosa non facilmente digeribile. Prendetela come un'affermazione politicamente poco corretta, ma questa è la sostanza dei fatti.

Da una parte, ci chiedono di semplificare, eliminare le norme, autocertificare, tutto ciò che può semplificare la vita, indubbiamente ormai insostenibile, di una famiglia o di un operatore economico o di un'azienda. Il pomeriggio avviene il contrario, perché si vogliono controlli, anche incrociati e più severi (sulla sicurezza del lavoro, sulla trasparenza degli appalti, sulle questioni ambientali): ogni sorta di giustissime finalità, che però comportano la eruttazione continua di nuove normative. Quindi, si tratta di fronteggiare questa duplice esigenza. Certo, l'ho detto all'inizio: sono un po' all'antica. Vorrei che invece di norme bastasse un clima morale della nostra società, poiché francamente è del tutto inconcepibile, la mia modestissima intelligenza, non solo che un funzionario si lasci corrompere ma che possa essere corrotto colui che ha chiesto la fiducia dei cittadini per via elettorale. Se è un mascalzone chi si fa corrompere e chi corrompe, chi si fa eleggere e poi si fa corrompere è un mascalzone due volte, e non troverei alcuna attenuante possibile e concepibile. Tuttavia, indubbiamente non indubbiamente non vorrei né sopravvalutare né sottovalutare questo testo. Non mi illudo che, varata questa normativa, saremo nella condizione di reprimere e prevenire, soprattutto, ogni forma di corruttela o di sviamento della pubblica amministrazione. Non mi illudo di questo. Però, tant'è: degli strumenti bisognerà pur metterli in campo. Al di là delle polemiche che sono state fatte, chiedo ai colleghi dell'opposizione: voterete contro cosa?

Voterete contro la costituzione, senza spese aggiuntive, non di un'autorità ma di un osservatorio a più voci e a più occhi sui fenomeni degli illeciti della pubblica amministrazione? Voterete contro il fatto che la trasparenza amministrativa diventi elemento costitutivo dei livelli essenziali delle prestazioni? Voterete contro l'obbligo della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni di tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi sensibili, degli appalti, dei concorsi? Vi chiedo, onorevoli senatori di opposizione: qual è qual è l'unico strumento col quale noi più sicuramente possiamo combattere i fenomeni di devianza o di malcostume se non quello dell'informazione la più ampia, la più capillare, la più accessibile da parte dei cittadini, degli utenti, di coloro che partecipano ad una gara, ad un concorso? La prima cosa è evidentemente aprire i cassetti, rendere accessibili le informazioni. Allora, lo sforzo che viene fatto in questo faticoso provvedimento è quello di prevedere un sistema di controlli incrociati e periodici e periodici e poi, di prevedere che il cosiddetto fallimento politico dia luogo anche a sanzioni severe nei confronti di chi è caduto in certi fenomeni deteriori o comunque ha fallito completamente gli obiettivi dei costi-benefici, rapportati a parametri oggettivi. Si dice che il rincrudimento delle pene è insufficiente.

perché non deve essere terrorismo penale ma deve essere adeguata la sanzione. La verità, onorevoli senatori, è che bisogna rendere effettive le pene, non semplicemente fare del terrorismo quantitativo, moltiplicando le pene stesse. Sono stati innalzati i minimi edittali. Non è un problema di agire sulla prescrizione, che è una norma di civiltà giuridica. Sono stati innalzati i minimi, e questo ha consentito di rendere più severe le sanzioni. Ma bisogna renderle effettive

perché si tratta di un tentativo che, se non esaurisce tutti i nostri doveri e potenzialità nel contrastare il malcostume, costituisce però sicuramente una linea, un fronte nettamente più avanzato rispetto all'attrezzatura giuridica di cui disponevamo fino a questo momento. Per queste ragioni, salvo valutare le proposte emendative, credo di poter esprimere a nome del mio Gruppo una valutazione complessivamente assai favorevole.

Signora Presidente, il disegno di legge che stiamo esaminando, trasmesso alla Presidenza il 4 maggio 2010, è stato oggetto di un'attenta considerazione in Commissione,

Colleghi, per cortesia. che ha registrato in Commissione pareri del Governo su emendamenti; anzi, su alcuni vi erano richieste di riformulazione,

Credo che tutti però dovremmo fare un salto di qualità nel dibattito, perché il fenomeno della corruzione

da parte dei cittadini e di coloro che operano nei settori maggiormente esposti che vi è un disvalore, generalmente condiviso dalle forze politiche

ma anche di coloro che si muovono nell'area della cosiddetta *border line* di raccomandazioni, di possibilità di incidenza sull'attività della pubblica amministrazione.

tali da garantire la trasparenza nell'attività della pubblica amministrazione, rendendo residuale la sanzione penale per comportamenti

Capi, i tre filoni cui ho appena accennato della prevenzione generale, dei controlli mirati e delle sanzioni specifiche. Vorrei solo fare un richiamo all'intervento del senatore Benedetti Valentini, proprio a proposito di sanzioni. Tutti siamo consapevoli che l'aumento della gravità della sanzione penale in sé non sempre è accompagnato da maggiore efficacia (anzi, molte volte, quando la pena è talmente alta da non essere percepita come giusta dal complesso dei cittadini abbiamo una situazione inversa, cioè non vi è quella capacità di deterrenza, proprio perché la norma non viene percepita come giusta e coerente con la finalità che persegue). La prevenzione del fenomeno di corruzione, di cui si occupa la prima parte del disegno di legge, che introduce una serie di misure, si ispira ad ad un mutamento culturale che introduce un disvalore complessivo volto a sanzionare

un danno alla credibilità dell'intero Paese e impedisce gli investimenti anche dall'estero. È questa È questa la ragione per cui il Governo si è mosso su una linea. Credo che, al di là della battaglia politica e della contrapposizione tra maggioranza e opposizione, dovremmo essere tutti consapevoli

si riuscirà a dare molto di più: una risposta coerente alla domanda di trasparenza che proviene dalla generalità dei cittadini. tutte le iniziative di prevenzione generale sono volte a dare risposta a questa domanda di trasparenza, una domanda che trova un'indicazione specifica nel Piano nazionale anticorruzione, che non è un invenzione, se volete, del Governo nel disegno di legge che è stato presentato una delle richieste degli Stati del Gruppo anticorruzione che fanno parte del GRECO. Questo Piano nazionale anticorruzione si connota anche per una rete nazionale anticorruzione composta dai referenti di ciascuna pubblica amministrazione, con il compito di fornire al Dipartimento della funzione pubblica elementi per la valutazione di idoneità degli strumenti adottati. alla conoscenza dei procedimenti amministrativi e alla possibilità per i cittadini di attuare un controllo generale che

e contempla controlli che devono funzionare perché il sistema democratico funzioni: da quello dell'opinione pubblica, della generalità dei cittadini, a controlli specifici cui sono deputati

oppure quando vi è la capacità del reo o di colui che devia di superare i controlli, riuscendo quindi ad ottenere lo stesso una devianza dell'azione della pubblica amministrazione. Se siamo convinti di questo, allora tutto il capitolo della prevenzione generale è l'indicazione sia di una serie di strumenti di trasparenza dell'attività amministrativa sia della possibilità di conoscenza da parte dei cittadini degli atti della pubblica amministrazione. Badate che solo attraverso quello che viene indicato con riguardo alla posta elettronica certificata, alla possibilità di controllo, alla pubblicità delle gare,

chi non è stato in grado di controllare la spesa pubblica o di avere un'attività amministrativa coerente con i principi di legalità, da un lato, e con i piani di compatibilità finanziaria, dall'altro, tale da non tale da non poter essere ricandidato alle successive elezioni. Questa disciplina si connota con una specifica norma sull'ineleggibilità ed incandidabilità alle cariche non livello degli enti locali, ma anche di deputato e senatore. Ciò determina un complesso di norme che si connota per una specifica capacità di controllo dell'azione della pubblica amministrazione.

Rispetto alla Convenzione di Strasburgo, di cui ieri è stata proposta in Commissione la ratifica, eravamo già d'accordo, maggioranza e opposizione.

io non ho criticato alcuni emendamenti che non accetto non dal punto di vista del Governo, ma da un punto di vista logico (ne abbiamo parlato anche in Commissione). pertanto che sarebbe molto più giusto che anche l'opposizione prendesse atto di una volontà complessiva dell'intero Parlamento e che tutti insieme, Governo al Parlamento, in modo che essa sia percepita come una corale e unanime azione della politica. Perché solo se l'azione della politica generale è percepita come tale dai cittadini potremo ottenere forse qualche successo nella lotta alla corruzione.

della deviazione rispetto alla corretta pubblica amministrazione. Ed è su questa linea che credo il Governo si atterrà nel dare i pareri ai singoli emendamenti, con l'auspicio che vi sia anche dall'opposizione, oltre che dalla maggioranza,

il quadro complessivo delle iniziative assunte dal Governo in materia di contrasto alla corruzione si è comunque sviluppato ed arricchito di una serie di episodi che giova ricordare, anche perché alcuni riguardano questa medesima legge.

grazie all'articolo 44 del decreto legislativo n. 235 del 2010, è stato stralciato perché le disposizioni contenute in quell'articolo riguardanti la disciplina della Banca dati nazionale dei contratti pubblici sono passate in quel decreto legislativo. Allo stesso modo è successo con l'articolo 4, le cui norme oggi ritroviamo nel decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. L'articolo 5, quello che prevedeva nel disegno di legge originario l'elenco dei fornitori e delle imprese di subappalto,

Oltre a questi elementi che riguardavano proprio la legge e che quindi, essendo inseriti nei decreti, verranno discussi altrove, anche se vanno considerati nella discussione che stiamo facendo, ci sono altre misure che sono stati assunte dal Governo, tra gli altri anche talune di natura finanziaria. Nell'ultima legge finanziaria abbiamo appostato 2 milioni di euro che serviranno, una volta approvato questo provvedimento, ad aiutare le Regioni con degli accordi di programma a trasferire in sede regionale alcune delle misure sia di semplificazione che di trasparenza e di contrasto alla corruzione. In altri momenti abbiamo assunto altre decisioni che sono comunque importanti sul fronte della lotta alla corruzione, ma che non sono invece riferibili a questa legge. In particolare nel maggio 2010 c'è stata l'approvazione della disposizione tributaria e finanziaria in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali; c'è stata la già ricordata decisione in finanziaria di stanziare questi 2 milioni di euro; nel settembre 2010, nell'Aula del Senato, è stato approvato il disegno di legge che ratifica la convenzione del Consiglio d'Europa contro la corruzione civile. credo che dovremmo leggere il provvedimento in esame in questo contesto, nella complessità dei provvedimenti che fin qui sono stati assunti. È ovvio che si tratta - come sempre accade quando si prende un'iniziativa di questa portata, che evidentemente ha anche dei caratteri innovativi - di un disegno non solo perfettibile, ma che è ben lungi dall'esaurire l'intera materia delle politiche di contrasto alla corruzione. Tuttavia, credo di aver colto nel dibattito alcuni segni contraddittori che, a mio avviso, è sbagliato trasmettere anche in termini di comunicazione fuori da quest'Aula. La decisione di affrettare - come ha voluto la Conferenza dei Capigruppo - la discussione prima dell'esame in Commissione degli emendamenti, sui quali era già stato reso il parere del Governo, è evidente che denuncia la convinzione comune di tutti i Gruppi, maggioranza ed opposizione, che sia importante approvare questo disegno di legge, altrimenti non capisco per quale ragione ne abbiamo fatto oggetto di un dibattito anche pubblico sui tempi dell'approvazione. Quando poi si coglie nel dibattito un depotenziamento o una banalizzazione dei contenuti di questo provvedimento, credo non si renda un buon servizio alla qualità del nostro dibattito. Ci sono tutti gli aspetti che ha già ricordato il collega Caliendo, a cominciare da quello dell'inasprimento delle pene che già è discuteremo, nel corso dell'esame degli emendamenti, se è il caso di rafforzarlo o meno. Ci sono iniziative importanti che raccolgono un'esigenza emersa anche nel dibattito della Commissione me, è stato un po' più ricco di come è stato reso in Aula), che sembrano trovare ampia condivisione. Ora si tratta di migliorare questo testo, ma ritengo sia molto importante che una serie di decisioni e di norme finalmente entrino nel nostro ordinamento: per aiutarci a fare cosa? La mia convinzione, che è soprattutto di natura culturale, è che la corruzione in Italia sia efficacemente contrastata sul piano della repressione, assai meno sul piano della prevenzione. La corruzione è un qualcosa che assomiglia vagamente a quei passaggi stretti che, nell'Età di nell'Età di mezzo, vedevano prosperare delle persone che indebitamente chiedevano tributi, facevano i passatori: dovunque si stringeva un passo, c'era qualche malintenzionato che riusciva a pretendere un tributo non dovuto. Noi abbiamo molti di questi passi stretti nella nostra burocrazia; e ovunque c'è poca trasparenza, ovunque c'è troppa discrezionalità, ovunque c'è una strettoia, la corruzione è un'eventualità latente, è un elemento che può diventare persino quasi funzionale rispetto a delle aspettative, soprattutto in aree e in regioni che sono fortemente inquinate dalla malavita e dalla criminalità organizzata. Questo provvedimento, insieme a tante altre leggi, insieme alle disposizioni che stiamo tentando di mettere in campo in materia di semplificazione e di trasparenza, serve ad allargare questi passi. Questo, a mio avviso, è il tema sul quale il nostro Paese è più indietro. L'efficacia delle politiche di contrasto di contrasto in sede repressiva da parte della magistratura, non fosse altro che per l'obbligatorietà dell'azione penale, non fosse altro che per i risultati che oltretutto vengono colti nel contrasto alla corruzione, è probabilmente superiore rispetto ad altri Paesi. L'eccesso di discrezionalità, che crea una burocrazia ancora pesante, ancora occhiuta, ancora in grado di creare enormi difficoltà a qualsiasi processo amministrativo: quello probabilmente è il fronte e il settore su cui dobbiamo intervenire. Questa legge non ha l'ambizione di realizzare tutti gli interventi possibili in questa materia, però certamente apre una strada e apre delle possibilità

Il provvedimento in esame è rimasto circa un anno in Commissione. Questo ci ha fatto assai dubitare del fatto che lo si riuscisse a disancorare dalle pastoie di un ritardo, di un remorare che non trovava giustificazione, rispetto all'urgenza e alla questione. In ogni caso, sottosegretario Augello, questa è l'Aula del Senato, il luogo è qui, ed è giusto che si svolga una discussione la più chiara possibile. Ora a nessuno di noi ovviamente sfugge, anzi abbiamo assolutamente presente che la questione della lotta alla corruzione non si esaurisce in un profilo. Non si esaurisce certamente nel profilo della repressione penale, come ha detto poc'anzi il sottosegretario Caliendo, sebbene essa abbia nel nostro nel nostro ordinamento una serie di profili che vanno guardati con grandissima attenzione e che non ineriscono soltanto all'innalzamento della pena - per esempio - piuttosto che alla possibilità di estendere la confisca anche ai proventi della corruzione, secondo modalità e con istituti che il nostro ordinamento già conosce. Ovviamente deve tener conto di un quadro complessivo anche processuale che oggi rende assai difficile un esito regolare dei processi per corruzione e che andrebbe riguardato rispetto all'importanza che annettiamo a questo profilo di illegalità. C'è poi un profilo economico. É quello - io credo - che più di ogni altro dovrebbe interessarci. Il sottosegretario Augello ha già fatto riferimento ad alcune norme che sono state introdotte. Nello stesso tempo, però, con grande chiarezza - l'ho apprezzato ha detto che non è soltanto il profilo della repressione quello che può aiutarci. C'è un profilo di prevenzione che assume in questo Paese, in questa fase, nella crisi economica e finanziaria grave del Paese un aspetto particolare. Non abbiamo più bisogno di leggere *report* che vengono da agenzie internazionali o da istituzioni italiane per sapere quanto la corruzione costa alle famiglie, alle imprese, allo Stato; quanto danno essa arreca al regolare funzionamento del mercato; quanto influisca sulla libera concorrenza. Cioè su tre pilastri, su tre questioni che sono centrali e sui quali il Governo dice di voler scommettere per il rilancio del Paese. Peraltro, proprio in questi giorni, la Commissaria per la giustizia è tornata su questo tema con grande forza strigliando - come si dice in linguaggio giornalistico - i 27 per

Anche se volessimo guardarlo soltanto da questo punto di vista, il testo che noi stiamo discutendo non è in linea con gli impegni che l'Italia ha assunto sulla base della Convenzione ONU,

ciò, in una situazione nella quale, al di là di chi sia il Presidente del Consiglio di questo Paese, sottosegretario Caliendo, è ovvio che ciò rappresenta una commistione che è impossibile da sciogliere. La stessa rete anticorruzione che sta dentro la pubblica amministrazione può essere un meccanismo di

Quello che vorrei evitare è che questa discussione diventasse una discussione nella quale dietro un adempimento formale di obblighi che il nostro Paese ha assunto si nasconda la volontà di non fare fino in fondo chiarezza e di non fare fino in fondo il nostro dovere. solo questo: una buona legge sulla corruzione, parziale come dite voi, perché non riusciremo a coprire l'intero arco delle questioni (c'è anche un capitolo di cui non si parla mai, che è il conflitto di interessi), ma una discussione vera. Se questo è lo spirito con il quale il Governo si mette a discutere di questo tema senza alibi, lo possiamo fare: l'Aula ne è la sede, e noi siamo prontissimi a farlo.

Presidente, colleghi, membri del Governo, l'Italia dei Valori ha tenuto a spingere, come altri Gruppi di opposizione, perché avviassimo una seria, serena e approfondita discussione del disegno di legge anticorruzione. È evidente - e mi rivolgo innanzitutto al sottosegretario Caliendo quando si affronta un problema così grave come quello della corruzione e, in special modo, della corruzione nella pubblica amministrazione, tutti noi, Governo *in primis*, dobbiamo farlo con spirito aperto, con cuore franco e con mente libera da qualsiasi forma di condizionamento, partendo dai dati reali che organi dello Stato, e mi riferisco in particolar modo alla Corte dei conti, ogni anno vieppiù sottolineano, facendo emergere le circostanze particolari in cui questo Paese si dibatte. che viene sovrastato da una corruzione sanguisuga, che sottrae risorse importanti ad un Paese che è in difficoltà socioeconomica, che cerca di dibattersi per superare la crisi partendo anche dalla riforma fiscale. Una buona legge anticorruzione serve anche a questo.

evitando concetti vuoti, ma andando al cuore del problema. Noi ci auguriamo, anche se fino ad oggi non abbiamo visto una volontà in tal senso, che questo si faccia. Altrimenti il Paese saprà che approverete una riforma anticorruzione che avrà lo stesso effetto di un'acqua fresca - neppure minerale - sparsa sul terreno.

di una approvazione burocratica di un testo, senza alcun apporto da parte delle opposizioni che attenga a questioni specifiche di merito,

l'attività delle pubbliche amministrazioni contro la corruzione. Ebbene, se questa è l'impostazione che il Governo e la maggioranza vogliono dare ai nostri lavori, certamente non potranno avere da parte nostra sconti rispetto all'esame del testo. Credo che invece bisognerà tener conto di tutta una serie di proposte che vengono dall'opposizione. Capisco che sono scomode, ma penso siano assolutamente utili, e su queste mi auguro vi sia la possibilità di un confronto serio in quest'Aula, e non solo per dire che abbiamo fatto finta di approvare un provvedimento anticorruzione.

intervengo per dire che la posizione del nostro Gruppo è molto chiara: riteniamo opportuno procedere nella discussione del disegno di legge, che peraltro risale ad un'iniziativa del Governo;

lascia liberi gli Stati. È quindi importante la valutazione del Parlamento ed anche del Governo sul recepimento di questa o quella norma nell'ordinamento penale, non essendovi un travaso momento che alcune norme possono essere compatibili con la nostra tradizione ed il nostro ordinamento penale, ed altre devono essere armonizzate all'ordinamento esistente. Riteniamo quindi

per l'entrata in vigore, che saranno effettuate le valutazioni per l'armonizzazione delle norme che la ratifica invita a fare nel nostro ordinamento penale - ad implementare la legislazione anticorruzione con ulteriori interventi. la disponibilità nostra, testimoniata anche dal voto favorevole di ieri nelle Commissioni, non deve servire a bloccare l'*iter* legislativo di questo provvedimento, dove liberamente il Parlamento si confronterà sugli emendamenti presentati.

non sarebbe una scelta positiva ed opportuna: lo consideriamo un lavoro importante, che sarà aperto agli ulteriori stimoli e contributi che l'entrata in vigore di intese internazionali proporrà, tenendo conto delle nostre tradizioni giuridiche, del nostro ordinamento, dei margini di discrezionalità che la stessa Convenzione di Strasburgo

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo e considerato che: - gli articoli 7 e 8 - nel novellare diverse disposizioni del testo unico leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs n. 267 del 2000) - intervengono in maniera incisiva sulla disciplina contabile degli enti locali e sul relativo sistema di controlli; - i predetti articoli 7 e 8 sono peraltro identici agli articoli 24

di dare luogo ad una produzione legislativa disorganica e del tutto disallineata rispetto al processo di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili previsto sia dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale sia dalla legge n. 196 del 2009 sulla contabilità pubblica; - a quest'ultimo riguardo, va ricordato che la Commissione sta esaminando l'atto del Governo n. ("disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi"), attuativo di una delega contenuta nella legge n. 42 del 2009, e ha già espresso il proprio parere sull'atto del Governo n. 359 (''disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili"), attuativo di una delega recata dalla legge n. 196 del 2009; esprime parere non ostativo sul testo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano soppressi gli articoli 7 e 8; osserva inoltre la necessità che, qualora nel testo siano presenti disposizioni riferite alla contabilità degli enti locali, l'Assemblea, in sede di approvazione del provvedimento, tenga conto delle premesse del parere. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere non ostativo, ad eccezione che sugli emendamenti 1.7, 2.11, 2.254,

fino alla fine del comma), 3.4, 11.0.3, 12.0.18 (limitatamente al comma 13), 1.200/2, 6.0.254 (limitatamente al comma 4) e 7.255 sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In relazione all'emendamento 1.200, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima disposizione costituzionale, alla soppressione del comma 3 e all'inserimento di una clausola clausola d'invarianza che escluda spettanze di ogni natura per i membri del Comitato. Esprime, poi, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria, sugli emendamenti 1.0.250, 3.253, 5.252 e 5.0.250. Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.3 e 3.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, riferiti agli articoli da 1 a 7. È rinviato l'esame degli altri emendamenti, a partire da quelli aggiuntivi all'articolo 7». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo a partire da quelli aggiuntivi all'articolo 7, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 7.0.251, 7.0.252, 8.250, 8.251, 8.0.1 e 8.0.250, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 7.0.254 e 12.251».

ma entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, dell'attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441, per quanto riguarda le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di titolari di cariche direttive di determinati istituti ed enti pubblici

votazione con reiezione, che sarebbe francamente ingiustificata. Quindi, accoglierei la disponibilità del Governo ad esaminarlo successivamente, trattandosi di un ordine del giorno di portata generale,

dispositivo, che riguarda l'annullamento dei benefici di legge nei reati di tipo economico e contro la pubblica amministrazione, ha in questo testo una condizione, che è quella del risarcimento integrale del danno. Piuttosto che di vittima, probabilmente bisognerebbe parlare di soggetto passivo, di parte offesa, perché in realtà si tratta spesso della pubblica amministrazione. Francamente, con questa condizione, io credo che il Governo dovrebbe ripensare al suo giudizio negativo perché c'è il risarcimento del danno che condiziona la possibile concessione delle attenuanti generiche degli altri benefici di legge.

Presidente, sapevamo che l'ordine del giorno era al limite rispetto alla materia della discussione. Tuttavia non vorremmo che in queste decisioni mancasse una capacità di cogliere quanto sconcerto c'è purtroppo nell'opinione pubblica rispetto ad alcuni fenomeni che pure accadono. Quindi, capiamo le difficoltà ed accettiamo la decisione della Presidenza.

in particolare di appalti pubblici e quindi della pubblica amministrazione, l'estraneità alla materia. Nulla toglie che altri strumenti e altre iniziative possano portare all'attenzione del Governo e del Senato la vicenda in oggetto.

Presidente, non voglio entrare nel merito della valutazione della Presidenza, che è sovrana. Però, il tema sollevato dall'ordine del giorno riguarda anche e prevalentemente le competenze pubbliche in materia di calcio e di scommesse, sia con riferimento ai poteri che lo Stato e l'Amministrazione centrale hanno in questa materia dal punto di vista delle concessioni e quant'altro, sia dal punto di vista dei poteri di vigilanza e di controllo che la pubblica amministrazione e lo Stato esercitano anche sulla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che è un soggetto che ha una sua rilevanza di diritto pubblico. Anche in ragione dell'attualità della discussione, purtroppo, e dell'emergenza e dello spaccato anche di queste ore e di questi giorni, mi permetto timidamente di dire che se fosse possibile riconsiderare tale questione, potrebbe essere anche un segnale che noi diamo rispetto a fatti che certamente non fanno onore ad una parte minoritaria, anche del calcio italiano.

gli emendamenti presentati, la Presidenza ha ritenuto in primo luogo improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, cioè per estraneità alla materia, gli emendamenti gli emendamenti concernenti incarichi e retribuzioni di pubblici dipendenti, magistrati e notai in quanto non strettamente attinenti al contenuto proprio del disegno di legge in esame, che riguarda la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Sono pertanto improponibili gli emendamenti

2.0.2, 2.0.250, 2.0.4, 6.0.3, 6.0.250,

La Presidenza ha ritenuto altresì improponibili, ai sensi della medesima disposizione del Regolamento, gli emendamenti 2.0.251, 8.0.1, 8.0.250, 10.0.2, 10.0.5, 10.300, 11.6, 11.0.5, recanti disposizioni relative ad attività dei parlamentari o di Governo, estranei al contenuto del disegno di legge, alcuni dei quali presentano inoltre profili di incostituzionalità. Dichiaro infine improponibili per estraneità all'oggetto della discussione gli emendamenti 2.0.5, 2.0.6, 3.0.1, 6.0.257, 8.0.251, 9.0.1,

12.0.17, 12.0.16, 12.0.100 e 12.0.18, relativi a modifiche di impianto generale al codice di procedura penale o a misure di natura fiscale e di razionalizzazione della spesa pubblica. Presidente, intervengo su questa declaratoria di improponibilità di numerosi emendamenti per esporre il punto di vista del nostro Gruppo e

principio condiviso e consolidato - da ultimo con il pronunciamo autorevolissimo del Presidente della Repubblica sul "milleproroghe", nei termini che conosciamo tutti relativamente ai decreti‑legge non viene in considerazione soltanto il tema della estraneità alla materia contenuta nel provvedimento legislativo, ma anche quello relativo alla funzione propria dello strumento legislativo e quindi ai presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione. Per i disegni di legge sappiamo invece tutti che i criteri di ammissibilità o di proponibilità, come vogliamo chiamarli, sono esattamente quelli previsti all'articolo 97, comma 1, del Regolamento e sono stati sempre adottati in modo abbastanza elastico. Ma io non invoco alcuna elasticità, quanto piuttosto una corretta applicazione di questa norma regolamentare.

(2.0.4, 6.0.3, 6.0.250, 6.0.251, 6.0.252 e 6.0.253) che riguardano gli incarichi extragiudiziari dei magistrati di tutte le magistrature ed i relativi compensi. Sono emendamenti presentati da molti Gruppi, non solo di opposizione, e che riguardano anche il tema delicatissimo, più volte discusso in questi anni, della incompatibilità dei magistrati rispetto alla partecipazione ai collegi arbitrali arbitrali o alle attività di collaudo delle opere pubbliche. qual è la ragione per la quale la Presidenza ha ritenuto non esattamente conferenti questi argomenti rispetto all'oggetto dell'articolato, questo tema, quello cioè della garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura e dei magistrati rispetto ad attività che hanno a che fare con l'assetto degli interessi dei privati e delle imprese nella gestione degli appalti pubblici e delle opere pubbliche, ha assolutamente a che fare con la materia che stiamo discutendo, cioè quella della prevenzione e della repressione, non soltanto della corruzione, ma dell'illegalità diffusa nella pubblica amministrazione. Non c'è alcun dubbio che i magistrati contabili piuttosto che amministrativi chiamati a esercitare la funzione di arbitro o di collaudatore di un'opera pubblica si collocano in una posizione, diciamo così, ambigua, di potenziale conflitto: ne abbiamo discusso molte volte. Come si fa a non ritenere compatibile e coerente con l'oggetto del provvedimento una materia così importante e così delicata quale quella di cui stiamo discutendo? In secondo

di vario genere, che non siano l'arbitrato e i collaudi, prevista nell'emendamento 6.0.254, così come in altri due emendamenti sempre in questa materia, il 6.0.5 e il 6.0.256, riguarda anche qui la tutela tutela della garanzia di imparzialità dei consiglieri di Stato muniti di funzione consultiva che - come propone l'emendamento - devono avere una funzione esclusiva per un periodo determinato di tempo. È evidente che la non esclusività della funzione consultiva di un consigliere di Stato pone i medesimi problemi a cui mi riferivo prima,

di deputati e senatori, nonché dei loro coniugi e figli. Non c'è alcun dubbio che il controllo della consistenza patrimoniale all'inizio, nel corso e alla fine del mandato dei parlamentari e dei rispettivi familiari abbia un rilevo

il tema dell'incandidabilità degli amministratori locali in rapporto alla commissione di reati di corruzione o comunque

oggetto del disegno di legge è fuori discussione. Lo stesso discorso vale per gli

in particolare nell'ultimo anno, e non solo. Questa norma consente di dichiarare «grande evento» - con tutte le conseguenze in ordine agli affidamenti in deroga degli appalti dei servizi e delle forniture pubbliche - una molteplicità di iniziative,

al sistema di affidamento degli appalti in deroga, sono esattamente quelli che originarono quell'ondata di arresti e indagini che hanno riguardato il mondo della Protezione civile e dintorni, a seguito del quale il Governo decise di presentare questo disegno di legge.

Parimenti, si dichiara improponibile l'introduzione del controllo preventivo della Corte dei conti sugli affidamenti in deroga. Come si fa? Ricordo che anche nel milleproroghe è stata introdotta una norma di questo tipo, un controllo successivo. Si può essere d'accordo o meno, ma anche questo tema riguarda indiscutibilmente la materia che stiamo trattando. In conclusione, signora Presidente, la prego di invitare il Presidente del Senato a rivalutare seriamente la declaratoria di improponibilità di tutti questi sottolineando che ove noi escludessimo dalla sola discussione il tema che riguarda le magistrature e il regime di incompatibilità, i parlamentari ed il regime di incompatibilità, la dichiarazione

desidero far presente che, come è noto, questo provvedimento è giunto all'esame dell'Aula senza mandato al relatore poiché le Commissioni riunite non hanno potuto completarne dovendo ancora esaminare e votare 200 emendamenti il giorno in cui è stato stabilito che il provvedimento approdasse in Aula. Ma l'*iter* del lavoro in Commissione è stato illustrato ieri dal presidente Berselli. Per questa ragione, e non per lassismo,

all'esame in 1a Commissione di provvedimenti autonomi - e che ciò avrebbe potuto essere motivo di inammissibilità. Non mi permetto - ripeto - di entrare nel merito delle decisioni e delle prerogative della Presidenza, però mi interessava

il segnale e lo spirito con cui si avvia questo percorso di lotta senza indugi alla corruzione, trovano un primo ostacolo nel fatto che venga dichiarata improponibile la sola prospettazione di inopportunità all'assunzione di incarichi di Governo di persone rinviate a giudizio per delitti contro la pubblica amministrazione. non stiamo anticipando i giudizi, ma se dobbiamo dire al Paese qualcosa, non prevedere il rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione quale motivo di inopportunità per l'assunzione dell'incarico di Governo ritengo non sia un messaggio che vada nella direzione auspicata da tutta l'Aula. Peraltro, prevediamo i casi di ineleggibilità per le condanne: qui stiamo parlando di inopportunità a ricoprire alcuni incarichi qualora si sia sotto processo per reati contro la pubblica amministrazione.

sul fallimento politico dei Comuni che siano in una fase di dissesto economico. economico. Mentre irrigidiamo legittimamente la nostra attenzione verso i Comuni, continuiamo a mantenere nel nostro sistema una depenalizzazione di fatto del falso in bilancio che continua a dare la possibilità per le società di creare

per poi fare operazioni finalizzate alla corruzione. È ovvio che, nel momento in cui con ampio spettro dobbiamo prevenire come ha evidenziato il Governo, l'attività di prevenzione è anche quella che riguarda la trasparenza dei bilanci delle società e quindi l'impossibilità, sanzionata penalmente e non depenalizzata, di costituire fondi neri per il pagamento dei prezzi corruttivi. Quindi, ritengo che l'onorevole Presidenza possa riesaminare tale decisione consentendoci di affrontare anche i temi che si inseriscono in questa comunicazione all'universo, e in particolare al popolo italiano, della crociata che stiamo avviando questa mattina.

Nel frattempo, come consuetudine, continuo a dare la parola sulle questioni attinenti all'ordine dei lavori a un senatore per Gruppo. Gruppo. Ovviamente, in attesa della decisione del Presidente, continuiamo i nostri lavori sull'articolo 1, che non è controverso, e sugli articoli e sugli emendamenti che non sono controversi, rimanendo inteso che in ogni caso

forse la prossima volta sarebbe opportuno avere a disposizione in Aula l'elenco degli emendamenti, in maniera tale che il nostro lavoro si possa svolgere con maggiore celerità.

in un provvedimento in cui si parla di disposizioni per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione non provare a regolamentare quel crinale fra i la rappresentanza degli interessi è legittima e quelli in cui è illegittima mi spinge a chiederle se si può ripensare

stanno al limite fra la questione procedurale-regolamentare ed una valutazione del merito del contenuto dell'emendamento. Ora, proprio perché non è stato possibile svolgere un lavoro preliminare nelle Commissioni di merito e non essendo noi accompagnati da un relatore nell'esame del provvedimento, il rischio è che la Presidenza diventi relatore di fatto di questo provvedimento

e le norme internazionali vigenti in Italia, segnalati già nel corso della discussione di ieri, segnalo come questo articolo 1, tra l'altro riscritto dal relatore e riproposto per certi versi in maniera più grave rispetto alle previsioni iniziali del testo,

della Convenzione ONU del 2003. In particolare, questo disegno di legge governativo contrasta con le norme ONU in materia di estensione delle fattispecie di reato (anche al settore privato), di poteri e strumenti di indagine alla polizia giudiziaria e alla magistratura, di misure di prevenzione adeguate ad affrontare il fenomeno corruttivo, di trasparenza nel settore degli appalti pubblici e della finanza pubblica, di misure antiriciclaggio, di termini per la prescrizione (termini che il testo ONU definisce necessariamente «lunghi», confisca dei beni, di cooperazione tra organismi di indagine (anche di *intelligence*), di inopponibilità del segreto bancario. bancario. Aggiungo che questo disegno di legge governativo contrasta pure con le analoghe norme che si trovano inserite nella Convenzione di Strasburgo del 1999, approvata il 7 giugno scorso, cioè ieri, all'unanimità dalle Commissioni giustizia e affari esteri di questo Senato, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di cooperazione internazionale, corruzione privata, riciclaggio e protezione dei cosiddetti testimoni. Con riferimento ai due emendamenti 1.200/1 e 1.200/5 e all'emendamento 1.3 che devo illustrare ora, rilevo un altro punto rilevante e specifico di contrasto con le citate Convenzioni internazionali, e in particolare con quella dell'ONU del 2003. Convenzione dell'ONU, all'articolo 6, prevede l'istituzione di un organismo per la prevenzione della corruzione indipendente e «al riparo da ogni indebita influenza» (così viene detto letteralmente), organismo al quale vanno fornite altresì risorse materiali e personale specializzato. Ora, la previsione nell'emendamento di un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, peggiora tra l'altro quanto inizialmente aveva previsto lo stesso testo del Governo. Francamente si tratta di una previsione che ci fa

tanto più che esso, sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri, opera come Autorità nazionale anticorruzione, a norma dell'articolo 5 della Convenzione ONU. Francamente c'è da rimanere allibiti, senza parole, per due motivi fondamentali. Non mi soffermo sul motivo di di tipo personalistico, perché andare a raccontare in Italia e all'estero che in questo momento il Comitato sulla trasparenza, anticorruzione sarà presieduto dal presidente Berlusconi fa quantomeno ridere, se non ci prendono addirittura per matti. Ma, al di là dalla considerazione personalistica, vorrei dire che, da un punto di vista istituzionale, vanno garantiti tutti, in tutti i momenti storici, con qualsiasi tipo di Governo. La domanda è sempre la stessa: *quis custodiet custodes*? Per un motivo di trasparenza, di pulizia e di rispetto delle regole, noi proponiamo qualcosa di alternativo, utilizzando norme già vigenti nel nostro ordinamento. Noi chiediamo che venga sostituita a questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione già approvata nel 2009 da questo Parlamento, oppure che vengono restituiti i poteri all'Alto commissario anticorruzione, sempre previsto dalla Convenzione ONU del 2009. È una scelta che poniamo al Governo. Finisco illustrando sinteticamente cos'è questa Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Ricordo che essa è stata istituita

opera in posizione che viene definita di indipendenza di giudizio e di valutazione, in piena autonomia, ma ovviamente in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con i vari Ministri, e ha il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale. Tutto questo riguarda il comportamento dei pubblici amministratori.

procedurale, che contempla anche l'intervento delle Commissioni parlamentari competenti tramite un parere che viene espresso a maggioranza dei due terzi. Credo che questo aspetto fondamentale dell'autonomia e dell'indipendenza debba essere garantito. Invece, con la proposta del relatore

con un aggravamento delle situazioni in termini di autonomia e indipendenza. La nostra proposta è alternativa: chiediamo al Governo di scegliere questa Autorità indipendente tra quelle che già esistono, cioè tra la Commissione che ho citato e l'Alto commissario anticorruzione.

la Commissione bilancio prevede una preclusione all'emendamento del ripristino dell'Alto commissario per ragioni di spesa. Personalmente, sono convinta che la funzione dell'Alto commissario sarebbe preferibile.

consentirebbe anche di dare un occhio al settore privato, materia rispetto alla quale noi proponiamo specifiche disposizioni anche di carattere penale per adeguarci alla legislazione internazionale. In ogni caso, stiamo violando la Convenzione ONU sulla corruzione. Questa è pertanto la dimostrazione che ratifichiamo le Convenzioni che sottoscriviamo, ma lo facciamo con la riserva mentale di non rispettarle.

l'Alto commissario per la lotta alla corruzione, sulla sua efficacia, sulla sua funzione e sul suo ruolo. Diamo per scontato che presso la Presidenza del Consiglio sia utile istituire questo Comitato anticorruzione. Però, se ha senso l'istituzione di questo Comitato, è necessario che esso abbia anche i poteri per esercitare una funzione. Questa funzione è innanzitutto di vigilanza e di controllo su tutte le amministrazioni pubbliche, esercitando anche un potere sostituivo nel caso in cui queste amministrazioni

perché, tranne qualche conferenza e qualche produzione cartacea di natura sovrabbondante, non sarà nelle condizioni di incidere minimamente sul fenomeno corruttivo. Per tale ragione, con l'emendamento

non fare le carezze alle amministrazioni, ma di intervenire in profondità per verificare se si adeguano o meno alla normativa anticorruzione.

istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato di coordinamento, sostituendo un comma 1 del testo originario in cui questo Comitato non c'era. Inoltre, esso prevede l'istituzione dell'Osservatorio

la clausola di salvaguardia al termine del comma 1, che afferma che sono escluse spettanze di ogni natura per i membri del Comitato,

Signora Presidente, l'emendamento 1.253 è molto simile a quello del senatore D'Alia

presso la Presidenza del Consiglio, chiunque sia il Presidente del Consiglio, perché credo che una legge debba stabilire dei principi e non debba essere legata ad alcuna persona. sia comunque un soggetto utile, se non altro per intervenire, come già sosteneva il senatore D'Alia, rispetto alle inadempienze delle amministrazioni. mi piace sottolineare due altri nostri emendamenti, signora Presidente, perché forse sfuggono alla nostra attenzione i punti che potrebbero essere i più importanti, quelli che riguardano la burocrazia: è come se approvassimo le leggi esclusivamente in senso punitivo nei riguardi dei politici, senza guardare bene ciò che accade all'interno della burocrazia

per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori».

da inserire in tutte quante le amministrazioni, a partire dalle stesse amministrative comunali, dove le incrostazioni della burocrazia diverse volte procurano danni superiori a quelli che eventualmente possono procurare i politici. Per ultimo, ma di valenza etica fondamentale, illustro il nostro emendamento 1.200/7, con il quale si prevede che «Coloro che occupano cariche pubbliche o assumano pubblici impieghi, all'atto della assunzione devono giurare fedeltà alla Costituzione italiana». Noi riteniamo che questo sia un emendamento che certamente non costa niente a nessuno, ma che costa moltissimo in termini etici, perché se è vero che viviamo in una società che ormai è priva di qualsiasi valore etico di riferimento, è pur vero che ciascuno di noi anche attraverso una legge anticorruzione vorrebbe dare quantomeno un indirizzo a tutti quanti coloro che debbono assumersi la responsabilità a livello centrale e periferico, in tutte quante le pubbliche amministrazioni.

Io sono stata sia sindaco che consigliere regionale e ho potuto appurare di persona che cosa significano la forza ed il potere che la dirigenza assume nei confronti dei politici: se, infatti, i politici si alternano, loro restano

dei dirigenti sia assolutamente indispensabile per la politica amministrativa diretta. [LI

previa concessione delle attenuanti generiche: in punto di fatto, il Presidente del Consiglio è stato riconosciuto colpevole di corruzione, ma non gli è stata applicata la sanzione perché gli hanno concesso le attenuanti generiche. all'emendamento 1.5. Si introduce il criterio della rotazione; benissimo. Ma non si può vanificare

l'Alto commissariato - che è stata sciolta e oggi è un Dipartimento della funzione pubblica ad occuparsi delle politiche di contrasto alla corruzione. La legge agisce dunque per implementare le capacità di questo Dipartimento: di questo stiamo discutendo. Dobbiamo però ricordare che l'Alto commissariato dipendeva dalla Presidenza del Consiglio esattamente come le strutture di cui stiamo parlando in questo momento.

Tra l'altro, sui motivi dell'intervento che ha portato allo scioglimento dell'Alto commissariato hanno pesato anche alcuni problemi che riguardavano il rapporto tra costi e benefici. La struttura aveva alcuni costi, che non dipendevano da una sua cattiva gestione, ma proprio dai costi strutturali, come la sede

il percorso che abbiamo cercato di indicare e di motivare in Commissione indica che in questo momento abbiamo, in primo luogo, il problema di mettere in linea una strumentazione e per questo si parla del Comitato interministeriale. Nel quadro che ho cercato di dare all'inizio del dibattito, ho cercato anche di illustrare all'Assemblea quali e quanti interventi si muovono all'intero della pubblica amministrazione sotto la medesima etichetta di politica di contrasto alla corruzione. Quindi, in questo momento e in questa fase, il Governo ritiene che questa sia la strumentazione da mettere in campo per garantire la massima efficacia della politica di contrasto alla corruzione, che passi attraverso tutti i vari Dicasteri e che richiede evidentemente un coordinamento. Non sfuggo

portata in linea, mentre altre realtà sono più avanzate della nostra. Quindi, a questo punto del percorso, diversamente da quanto era accaduto con l'istituzione dell'Alto commissariato, che dipendeva comunque dalla Presidenza del Consiglio e non aveva autonomia, pensiamo che questa sia la strumentazione che deve essere portata all'attenzione del Parlamento.

2)/4, il parere è contrario perché il processo di coinvolgimento delle Regioni dovrà avvenire diversamente, non nel Comitato interministeriale ma attraverso una serie di accordi

questioni poste dal sottosegretario Augello. Qui non si mette in discussione la istituzione e la costituzione di un progetto e di un lavoro presso la Funzione pubblica o la Presidenza del Consiglio di coordinamento delle amministrazioni pubbliche nella lotta alla corruzione, nel migliorare le proprie prestazioni, quanto la mancanza - e questo credo sia un principio generale dell'ordinamento, almeno dei Paesi che conosciamo in democrazia - di una distinzione netta tra controllore e controllato. È per questo che stiamo insistendo nelle forme varie, attraverso gli emendamenti, rispetto a chi controlla

che dovrebbe essere affidato ad un'autorità indipendente. È su questo punto e con queste motivazioni che sono per noi fondamentali rispetto alla costituzione e all'avanzamento di questo provvedimento, che dichiaro il voto favorevole

Presidente, le posso far osservare che il Governo ha espresso un parere sull'emendamento 1.0.250, che però, essendo stato numerato diversamente, verrà discusso

Penso all'indagine sul Policlinico, alle varie indagini sugli ospedali in Calabria, alle indagini sull'università, all'istituzione del numero verde al quale si rivolgevano i cittadini. Appena insediato, questo Governo ha immediatamente chiuso l'ufficio, ricevendo il biasimo di tutta l'Europa, ragion per cui è stato riaperto alla svelta

Senatore De Angelis, di chi è quella scheda?

Senatore Asciutti, non è questo il problema. Il punto è che ci sono coloro che votano per quelli accanto e coloro che dove c'è la scheda non votano.

chiedo di sopprimere le parole finali «che costituisce ufficio dirigenziale di livello generale». Resta pertanto «il Dipartimento», e

l'espressione «specificano procedure appropriate per selezionare». Ricapitolando, la nuova formulazione dell'emendamento rispetto al testo stampato prevede la clausola di invarianza al termine del comma 1, già precedentemente

Il tema centrale è sempre lo Non possiamo pensare che il contrasto alla corruzione lo si faccia con una struttura di coordinamento e non lo si faccia attraverso un'Autorità indipendente: lo ripeteremo per tutto l'andamento di questi lavori.

c'è una questione di fondo: non possiamo metter su un ennesimo pachiderma che non ha alcuna funzione efficace nella lotta alla corruzione

Gruppi parlamentari e dell'opposizione, si sono battuti per far calendarizzare questo provvedimento, confidando e sperando nella possibilità di trovare un testo condiviso anche con la maggioranza: fino ad ora ci

ricorderanno che l'Assemblea Costituente si occupò del tema del giuramento dei parlamentari alla Repubblica e alla Costituzione, e concluse che

di politiche di contrasto alla corruzione, abbiamo necessità di esaminare quali siano le possibilità di proseguire questa discussione, come pure gli effetti tecnici della bocciatura di questo articolo sulle altre previsioni della legge contenute negli articoli successivi. Ovviamente, dal momento che stiamo lavorando a braccio,

lo stesso *incipit* dell'intervento del sottosegretario Augello - l'essere caduto con l'articolo 1 il pilastro intorno al quale era costruito il disegno di legge - conduce, inevitabilmente, mi sia consentito dirlo in maniera molto

Il provvedimento è caduto nel suo asse principale, che noi consideravamo sbagliato. E non sarà sfuggito che è esattamente sull'articolo 1 che si era articolata la critica

Comunque, il Governo ha chiesto tempo fino alle ore 16. Noi, nel frattempo, ovviamente adotteremo le iniziative politiche che riteniamo di dover adottare, ma mi sembra che stiamo reggendo una finzione che non so a chi faccia bene. La verità è di fronte a noi: il provvedimento è caduto. Il Governo lo ritiri.

evidente che il Governo preliminarmente deve dire se condivide la posizione espressa dal Gruppo del Partito Democratico, ma deve riversare le sue opinioni nella Commissione e poi venire in Aula avendo valutato se ci sono le condizioni per chiudere l'esame di questo provvedimento o ripartire attraverso una riformulazione dell'articolo 1, dunque dell'impianto fondamentale della normativa. per la civiltà del rapporto tra Governo e Assemblea, tutto ciò si possa risolvere con una comunicazione del rappresentante del Governo all'Aula del Senato come una decisione unilaterale del Governo. Penso che ciò debba avvenire nella sede della Commissione, e qui si debba esercitare quella

a me dispiace, non voglio fare polemiche, però lei ricorderà che sia ieri che stamattina, sia sull'ordine dei lavori che all'inizio della discussione relativa all'esame degli emendamenti, avevamo chiesto che la maggioranza e il Governo si pronunciassero sulle proposte che venivano da parte dell'opposizione funzionali a modificare un testo presentato dal Governo, perché l'articolo 1 fa parte del disegno di legge, signor Sottosegretario, che reca come prima firma quella del Ministro della giustizia, l'onorevole Alfano, poi quelle dell'onorevole Maroni, dell'onorevole Bossi, dell'onorevole Calderoli al suo articolo 1 prevedeva una versione estremamente *soft*, leggera, inutile, inefficace sul piano della lotta alla corruzione, è stato bocciato dall'Aula. o voi non avete un'idea di come volete condurre la lotta alla corruzione nel Paese, e allora questo momento di riflessione serve a poco (ritirate quindi il disegno di legge o discutiamo dei nostri provvedimenti che sono abbinati a quello, nelle forme e secondo le procedure che prevede il Regolamento), oppure dovete dirci se intendete fare un accordo con le opposizioni su un testo che sia realmente utile ed efficace al contrasto e alla lotta alla criminalità, proposto voi è stato bocciato dall'Aula e dovete prenderne atto dal punto di vista politico; dovete prenderne atto perché non c'è una politica del Governo e della maggioranza su questa materia.

Presidente, colleghi, ritengo che il Governo e la maggioranza siano fortunati, siano fortunati, perché avremmo corso il rischio di affidare il coordinamento dell'anticorruzione a chi problemi di corruzione ne ha ancora in questo momento. Questa era la prima osservazione. Passo alla seconda osservazione. Questa mattina, nell'intervento che abbiamo fatto noi dell'opposizione, abbiamo dichiarato in modo chiaro chiaro che l'unica cosa di epocale che riuscite a fare è prendere in giro le opposizioni e il Paese. Questa volta le opposizioni vi hanno dimostrato che non ci stanno più; il Paese ve l'ha dimostrato qualche domenica fa, e continuerà

Signor Presidente, noi del Gruppo della Lega Nord riteniamo sia giusto dare tempo al Governo per valutare gli effetti della soppressione dell'articolo 1, votata in quest'Aula. dunque giusto attendere le ore 16 per fare le opportune valutazioni. Abbiamo letto dalle agenzie che le opposizioni hanno già indetto una conferenza stampa nel primo pomeriggio.

la proposta di istituire il Piano nazionale anticorruzione ed un apposito Osservatorio che sarebbe stato bene approvare nell'Aula del Senato, dato che l'effetto pratico è esattamente quello che

PdL).*Questo in punta di fatto. In punta di polemica politica, ovviamente, siamo pratici delle cose di mondo e comprendiamo che ciascuno può argomentare come ritiene. Il Governo ha bisogno di una pausa per verificare

articolo pone dei problemi di ordine politico, di ordine procedurale e di ordine regolamentare. Ma c'è una grande questione che riguarda sia la maggioranza che l'opposizione. Credo che abbiamo tutti il dovere di fare una riflessione aggiuntiva, oltre quella che dovrà fare il Governo, e riportare nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo la discussione ed il confronto per determinare l'utilità di questa settimana e per fare in modo che comunque il Parlamento, preso atto di quello che è accaduto, sia in grado, maggioranza e opposizione... FINOCCHIARO *(PD)*. C'è il testo Stavo dicendo, e quindi mi stavo rivolgendo anche alla senatrice Finocchiaro, che maggioranza e opposizione hanno entrambe il dovere, preso atto di quanto è accaduto, che si legge in termini chiari sul piano politico, regolamentare e procedurale, di utilizzare utilmente questa settimana per dare un segnale anticorruzione, un segnale da parte di tutte le forze politiche, cosa che è possibile ed è rimessa all'intelligenza della senatrice Finocchiaro e dei Capigruppo di maggioranza.

sono ostaggio di disservizi, di file chilometriche agli sportelli. L'amministratore delegato, appena riconfermato, l'ingegnere Sarmi, si è scusato per i disagi e i disservizi che ancora questa mattina sono stati registrati in tantissimi uffici postali ed ha aderito alla proposta di un tavolo di conciliazione, la quale era stata fatta da alcune associazioni dei consumatori. Questo tavolo si dovrebbe aprire domani, anche per valutare i risarcimenti dei danni inferti a tantissimi pensionati che hanno dovuto sorbirsi ore e ore di fila per disfunzione del sistema elettronico. Abbiamo appreso, signor Presidente, che nel 2005 Sarmi ha firmato il primo contratto a 12 milioni di euro per informatizzare gli uffici postali con il *software* della IBM. Lungo la strada i 12 milioni sono lievitati a 90 milioni ma, per vedere gli effetti di detta operazione, bisogna arrivare all'ottobre 2010. Al marzo di quest'anno, Sarmi, assistito dal capo della rete Bragazzi, assegna sempre all'IBM 150 milioni di euro con l'obiettivo di informatizzare, entro giugno, altri 10.000 uffici postali. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Stando ad indiscrezioni di stampa, la relativa gara di 150 milioni avrebbe visto un solo partecipante, l'IBM, il quale, per assegnarsi la commessa, avrebbe applicato alla sua offerta un gentile ribasso del 4 Adesso la nuova architettura è crollata. I tecnici di Armonk, sede canadese dell'IBM, stanno cercando di risolvere quello che, in una nota diffusa ieri, è stato definito in maniera troppo semplicistica un inconveniente al *software* in via di completa risoluzione. Signor Presidente, colleghi, i consumatori, i cittadini, i pensionati e le famiglie non possono continuare a pagare i disservizi

con le esigenze che pongo in quest'Aula. Ma bisogna capire che non se ne può più. I cittadini, e lo dimostreranno anche - ci auguriamo

la 4-05289, presentata insieme alla senatrice Poretti, alla quale anche la senatrice Carloni ha deciso di apporre la sua firma (ricordo che la senatrice Carloni è oggi a Parigi in missione). Entrambe hanno a che fare con i centri di identificazione ed espulsione: in particolare, la prima con il centro di identificazione ed espulsione di Santa Maria Capua Vetere. La seconda chiede informazioni circa i motivi per i quali non soltanto ai CIE, ma anche ai centri di assistenza per coloro che chiedono l'asilo, è stato proibito l'accesso alla stampa. La presenza di operatori dell'informazione, che in modo indipendente possono anche smentire le dichiarazioni che fanno non soltanto le forze dell'ordine e i trattenuti ma anche i parlamentari che visitano in queste ore i centri, è fondamentale. Lo dico - per esempio - perché stanotte, alle ore 3, ci è giunta notizia

tre visite del Ministero dell' interno. Siccome le cose si sanno, occorrerebbe rispondere in maniera formale, anche perché siamo in patente violazione, sistematica e continuata, dei diritti fondamentali di decine e decine di persone che non sono cittadini italiani. Nel caso di specie, si tratta di 96 cittadini tunisini trattenuti, contro tutte le norme vigenti, nazionali ed internazionali,

in un centro per l'identificazione e l'espulsione, dove non ci sono letti, tavoli, sedie, dove i bagni sono all'esterno della tenda, dove vengono trattenute le persone

Signor Presidente, l'intervento del senatore Lannutti a proposito dei disservizi

come tutti sappiamo, di eccellente livello, e che fa oggi i conti con nuove e moderne esigenze. Tuttavia, il tema probabilmente più urgente da focalizzare è quello che riguarda all'interno del servizio postale quella universalità che è un principio caro, che difendiamo, pur nel processo di liberalizzazione del servizio postale. Forse, all'interno di questo, un'ulteriore riflessione può e deve essere fatta riguardo l'affidamento e l'esternalizzazione di alcuni servizi

ai quali il servizio postale deve essere comunque garantito. Non dimentichiamo infine che da lì passa anche una parte della gestione di quel risparmio postale che è uno dei capisaldi capisaldi della solidità del sistema economico italiano. Rispettosi di questo, credo che sia giusto approfondire come mai ci si è trovati in questa situazione.

La pregherei di attivarsi in questo senso per mettere il Parlamento nelle condizioni di conoscere a fondo tutti gli aspetti che hanno riguardato questa vicenda. **Per Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia voce a quella del senatore Perduca. Nelle settimane scorse la Commissione per i diritti umani ha effettuato una missione